Signor Presidente, nell'interrogazione presentata il senatore Gramazio si riferisce, a partire da articoli di giornale, a fatti relativi alla città di Roma in relazione alla questione sfratti e ai ritardi relativi al contributo affitti. Per quanto riguarda la questione sfratti, si fa notare che la nobile azione operata dal prefetto Serra riguardo alla istituzione della commissione di graduazione degli sfratti è frutto di una possibilità data dalla legge 15 febbraio 2007, n. 9, al fine di trovare, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, forme di passaggio da casa a casa per gli sfrattati. Si segnala a tal fine che la citata commissione, ove istituita, ha il compito di graduare gli sfratti dei soggetti citati dalla legge, ovvero portatori di *handicap*, anziani, malati terminali, famiglie con figli a carico fiscalmente, purché con sentenza di sfratto per finita locazione e con reddito inferiore ai 27.000 euro, e dei soggetti con sfratto in esecuzione collocati utilmente in graduatoria. Si fa anche presente che nella Regione Lazio possono partecipare ai bandi per l'assegnazione di una casa popolare anche coloro con sfratto per morosità. Quindi, pur non avendo esplicitamente sospeso gli sfratti anche per le famiglie con sfratto per morosità, si è fornita alle prefetture una possibilità di graduare anche gli sfratti per morosità relativi a nuclei famigliari con condizioni di particolare disagio riconosciuto e certificato attraverso la presenza nelle graduatorie. Ci auguriamo che l'iniziativa intrapresa con grande sensibilità dal prefetto Serra sia da traino per analoghe iniziative da parte degli altri prefetti interessati. Come il senatore Gramazio sa, non è certo con le sospensioni degli sfratti che si garantisce il diritto alla casa ma attraverso una politica strutturale. Anche su questo versante la legge n. 9 del 2007 ha prodotto un primo rilevante risultato: proprio ieri il tavolo nazionale di concertazione sulle politiche abitative, istituito dalla citata legge, ha concluso i lavori ed ha elencato in un documento le indicazioni che dovranno essere alla base del piano nazionale sulla casa che entro sessanta giorni Governo e Conferenza unificata dovranno elaborare indicando a loro volta obiettivi e linee guida. Si tratta di un documento complesso e articolato che può essere la svolta da tempo auspicata nelle politiche abitative e sul quale il Governo intende impegnarsi ritenendo la questione abitativa una priorità. Appare evidente, da quanto affermato, che il Governo ha avviato un percorso che, sulla base dei programmi comunali e regionali, risponda a tutte le articolazioni dell'emergenza abitativa. Del resto, lo stesso Parlamento sarà chiamato ad esprimere un parere sul piano nazionale entro il prossimo 15 luglio. Per quanto riguarda il contributo affitto, effettivamente, e nell'immediato, è l'unica risposta di contrasto alla morosità ed è vero che sconta a tutt'oggi dei ritardi nei meccanismi di elargizione alle famiglie interessate e che ne hanno diritto. Non essendo solo un problema della Regione Lazio e del Comune di Roma, da una parte stiamo valutando e considerando la possibilità di aumentare le risorse disponibili per il contributo affitto, anche tenendo conto delle richieste del tavolo nazionale di concertazione sulle politiche abitative, e dall'altra il Ministero della solidarietà sociale intende discutere con gli altri Ministeri competenti, con le Regioni e l'ANCI la possibilità di intervenire sulle procedure per cercare di snellirle al fine di evitare che il contributo affitto arrivi con ritardi non comprensibili. Il nostro obiettivo è di avviare una politica abitativa che affronti strutturalmente la questione abitativa attraverso la riapertura di un dialogo e una concertazione con tutti i soggetti interessati e non in maniera emergenziale o attraverso alienazioni di patrimonio pubblico che hanno semmai peggiorato la situazione in essere, come fatto d'altronde dal precedente Governo.

Il buono casa non può essere solo un piccolo contributo: per queste famiglie il buono casa diventa un momento importante. Cioè, il buono casa pagato regolarmente permette

a garanzia di questi cittadini. Voglio ricordare che in una città grande come Roma il problema è pressante per l'amministrazione locale,

ovviamente rilevanza all'attività del CESI Ricerca S.p.A., che è uno dei centri nazionali più avanzati di ricerca nel settore elettrico. Proprio per consolidarne l'attività e consentire l'attribuzione delle risorse previste dal Fondo per la ricerca nel settore elettrico, a luglio del 2006 il Ministero ha dato indirizzi all'ENEA di procedere all'acquisizione del 51 per cento delle quote azionarie e di definire un piano strategico per la valorizzazione e il riposizionamento della società, con indicazione delle modalità e dei meccanismi di finanziamento delle attività, anche in aggiunta alle risorse disponibili sul Fondo per la ricerca di sistema elettrico, aspetto che assume un'importanza decisiva ai fini dello sviluppo futuro della struttura. Dopo l'approvazione da parte della Commissione europea-Direzione generale concorrenza, in data 20 dicembre 2006, del regime di finanziamento alle attività di ricerca e sviluppo nel settore elettrico che ha ritenuto «non aiuto di Stato» il finanziamento delle attività di ricerca a finalità pubblica - si sono avviate le attività di attuazione dei decreti ministeriali dell'8 e del 23 marzo 2006, allo scopo di arrivare rapidamente alla stipula dell'accordo di programma con CESI Ricerca S.p.A. per l'anno 2006 e alla predisposizione di un piano anche per l'anno 2007. I due decreti del 2006 sono stati, tuttavia, giudicati dagli organi di controllo una base giuridica inadeguata ed insufficiente a giustificare la legittimità degli accordi di programma. Pertanto, ferma restando la necessità che i soci definiscano una strategia di riposizionamento della società e che si lavori per riguadagnare i necessari margini di efficienza gestionale, il Ministero si impegna a promuovere nei prossimi giorni una soluzione in via normativa, che legittimi gli accordi di programma e consenta la definizione di impegni per il 2006 e per l'anno in corso.

POSSA *(FI)*. Ringrazio l'onorevole sottosegretario Gianni per la sua risposta, che tuttavia non mi soddisfa

del 23 marzo 2006 sono stati ritenuti una base giuridica non sufficiente per procedere all'accordo di programma con CESI Ricerca S.p.A. Ci vuole un anno

il Sottosegretario non ha riferito alcuna motivazione di queste incertezze giuridiche che minano l'applicabilità dei due decreti ministeriali dell'8 marzo 2006 e del 23 marzo 2006. Non ci si rende conto delle difficoltà che occorre superare e che comunque il Ministero si è impegnato a risolvere nei prossimi giorni. tuttavia oltre un anno alle spalle per valutare effettivamente se questi due decreti ministeriali del Ministero delle attività produttive avessero una base solida per poter procedere all'accordo di programma. Uno dei primari centri di ricerca italiani nel campo elettrico, in ambito pubblico sicuramente il numero uno,

il *deficit* del consuntivo 2006 non gli consente di raggiungere il *quorum* necessario per procedere finanziariamente e amministrativamente. Siamo in una situazione drammatica, signor Presidente, e devo dire che la risposta, pur animata evidentemente da buona volontà del Sottosegretario, e del Ministro ieri alla Camera, non

quattrini che sono a disposizione perché già prelevati, tramite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalla bolletta elettrica. Siamo al paradosso: abbiamo i fondi per finanziare la ricerca, abbiamo la struttura legislativa

mi dichiaro soddisfatto per la risposta. Ritengo tuttavia necessario sottolineare che, per evitare la messa in liquidazione della

dell'energia e dell'elettricità. per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, la società cooperativa Regione Campania 349 è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 23 novembre 1999 e sono stati nominati tre commissari liquidatori. Successivamente, nel 2000, a seguito della rinuncia all'incarico da parte dei tre commissari, è stato nominato un solo commissario liquidatore con decreto ministeriale del 28 dicembre 2000. Al momento della messa in liquidazione, il patrimonio immobiliare era costituito da 55 alloggi, completati e assegnati a soci ed occupanti senza titolo, nonché da beni immobili ancora da completare (negozi e sottotetti). Su detti beni l'istituto San Paolo di Torino (il cui credito ammontava ad oltre 30 miliardi di lire) aveva iniziato, già dall'anno 1992, azioni di esproprio immobiliare. Tutto il patrimonio immobiliare era stato realizzato su aree in ordine alle quali il Comune di Pollena Trocchia aveva concesso il diritto di superficie, mediante stipula di apposita convenzione. I beni edificati risultavano, quindi, di esclusiva proprietà della predetta cooperativa. Con delibera consiliare del 28 novembre 2001, il Comune di Pollena Trocchia dichiarò decaduta la convenzione, limitatamente agli interventi edilizi non realizzati o parzialmente realizzati. Erano assenti le condizioni per tutelare le ragioni economiche e sociali dei soci e degli occupanti, per chiudere la liquidazione attraverso l'adozione di un concordato articolo 214 della legge fallimentare). In particolare: i crediti privilegiati (rappresentati dagli istituti bancari) erano superiori ai 30 miliardi; i crediti chirografari erano superiori ai 2 miliardi (senza considerare i debiti della cooperativa nei confronti dei soci); i soggetti che avrebbero dovuto accollarsi la proposta erano i soli soci assegnatari (che risultavano essere 32), con una conseguente abnorme esposizione individuale, anche nell'eventualità (peraltro teorica) di una proposta di pagamento del solo 50 per cento dei crediti privilegiati per cento di quelli chirografari. Si è quindi intrapresa necessariamente la strada della vendita del patrimonio, sempre cercando di salvaguardare le ragioni dei soci e degli occupanti. È in tale ottica che venne, infatti, formulata una proposta transattiva, in accordo con i soci e gli occupanti, con un prezzo medio per alloggio di 100 milioni di lire. Furono in particolare previste due diverse fasce di prezzi: per i lotti 11 e 12 i soci assegnatari avrebbero dovuto versare 88 milioni di lire e gli occupanti senza titolo 125 milioni di lire, mentre per il lotto 50 i soci avrebbero dovuto versare 65 milioni di lire e gli occupanti 70 milioni di lire. I soci e gli occupanti sottoscrissero 33 proposte di acquisto; il commissario liquidatore formulò per iscritto la proposta, che venne accettata il 6 giugno 2001 dalla SIB spa, società di gestione dei crediti dell'istituto San Paolo di Torino che, nel frattempo, aveva ceduto i propri crediti. Successivamente, da parte di alcuni occupanti senza titolo che non avevano sottoscritto la proposta d'acquisto, fu avanzata la richiesta di sottoscrizione a condizione che l'importo da versare fosse ridotto da 125 a 100 milioni di lire. Il commissario liquidatore manifestò perplessità rilevando che le proposte di modifica dovevano, comunque, essere sottoposte al consiglio di amministrazione dell'istituto di credito. Alla fine del mese di giugno 2001 vennero notificati alla liquidazione sette atti stragiudiziali (ad istanza di 14 soci storici, 10 aspiranti soci delle mansarde e 10 aspiranti soci assegnatari, anche da parte di soggetti che avevano già sottoscritto la proposta di acquisto nell'ambito dell'accordo transattivo) nei quali si sosteneva che la cooperativa non poteva essere assoggettata a procedura fallimentare e che il relativo patrimonio, facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato, non poteva formare oggetto di vendita. Si cercò di organizzare un incontro chiarificatore presso il Ministero delle attività produttive, che però non ebbe luogo a seguito della mancata disponibilità all'incontro del rappresentante legale dei soci interessati. Nel 2001 l'autorità di vigilanza autorizzò il commissario liquidatore ad alienare, a trattativa privata, gli immobili di proprietà della liquidazione coatta amministrativa (ad eccezione del L'autorizzazione alla vendita sarebbe avvenuta in favore di alcune cooperative («Il Villaggio» e «Magnolia») che avevano formulato proposta cauzionata d'acquisto e si assumevano l'impegno a trasferire la proprietà degli immobili agli occupanti degli alloggi al prezzo già proposto ed accolto dalla predetta SIB (diverso, come ho già detto, a seconda che l'acquirente fosse socio della cooperativa od occupante senza titolo), purché la richiesta da parte degli interessati fosse esplicitata entro e non oltre il 15 novembre 2001. Dopo riunioni svoltesi presso il Ministero delle attività produttive e il Comune di Pollena Trocchia, nonché l'occupazione della casa comunale, è stato fissato un nuovo ultimo termine per l'esercizio dell'opzione all'acquisto al 18 maggio 2002. A novembre 2006 per i 55 alloggi completati ed occupati l'opzione all'acquisto è stata esercitata da 27 soggetti tra soci ed occupanti senza titolo (praticamente, dal 50 per cento degli stessi); per i restanti 28 sono in corso giudizi per il rilascio dell'immobile. Nell'anno in corso, presso le sedi del Ministero dello sviluppo economico e della Regione Campania si sono svolti due incontri, che mi hanno visto promotore,

Trocchia) interessate alla risoluzione delle problematiche riguardanti gli ex soci della cooperativa in oggetto e degli acquirenti degli alloggi. Nel corso dell'ultima riunione, tenutasi precisamente a Napoli, ho personalmente avanzato anche una proposta di mediazione, stessa riunione è emersa la volontà degli acquirenti di non aderire alla proposta di una ulteriore proroga di otto mesi per la esecutività degli sfratti.

e il Ministero per la chiarezza della cronistoria, che conferma in larga parte ciò che noi nell'interrogazione avevamo già significato, ma anche - l'ha ricordato lei stesso, signor Sottosegretario - il fatto che lei risponde conoscendo i fatti, in quanto ben due volte in

una storia grave che nega di fatto il diritto alla casa a soggetti che in cooperativa hanno tentato di contribuire, con il frutto del loro lavoro, ad esercitare un diritto costituzionale, di cui parlava prima

Non discuto, ovviamente, le procedure di esproprio da parte della banca, ma ritengo che il commissario liquidatore avrebbe dovuto tutelare maggiormente i soci truffati.

a stare su questo terreno. C'è un fatto che posso testimoniare personalmente, essendo stato eletto in quell'area: c'è una continua vendita di beni che hanno acquisito un valore perché, giustamente, il Comune di Pollena Trocchia ha un piano regolatore che non prevede molte altre occasioni. In primo luogo fatta una riflessione sulla funzione di vigilanza, che non può essere solo tecnica - sul piano formale è tutto a posto - ma a mio avviso avrebbe dovuto meglio comparare gli interessi, in particolare di coloro che, a torto o a ragione, si ritengono truffati. In secondo luogo, sicuramente c'è una grave responsabilità del Comune di Pollena Trocchia, che bene avrebbe potuto, in quanto concessore del diritto di superficie, condizionare

le infrastrutture*. In merito a quanto richiesto dal senatore Iovene nell'interrogazione a cui si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28 marzo 2007, la società Ferrovie dello Stato ha fatto conoscere che la vicenda della soppressione del passaggio a livello al chilometro 320+499 della linea Metaponto-Reggio Calabria ha avuto inizio nel 1988 quando, a seguito di accordi specifici, il Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, con delibera n. 88 del 28 novembre 1988, ha approvato il progetto delle opere sostitutive e la convenzione che regolava i rapporti tra le Ferrovie dello Stato ed il Comune per la realizzazione di un sottovia al chilometro 320+773 della stessa linea. La società Ferrovie dello Stato informa che i lavori, seppure appaltati, non ebbero inizio in quanto il Comune non ha mai messo a disposizione le aree necessarie per la loro realizzazione. In seguito, lo stesso Comune si è dichiarato interessato all'eliminazione del passaggio a livello in argomento a fronte della realizzazione di un nuovo sottovia al km 320+493, il cui progetto è stato approvato in data 30 aprile 1998 con delibera n. 15 del Consiglio comunale. La nuova convenzione regolante i rapporti derivanti dalla soppressione del passaggio a livello, approvata con delibera del Consiglio comunale n. 29 del 4 ottobre 2001, prevede che RFI realizzi le opere sostitutive e che il Comune metta a disposizione tutte le aree necessarie provvedendo allo spostamento dei sottoservizi interferenti con le opere stesse. A seguito di gara di appalto, i lavori sono stati aggiudicati in data 1° agosto 2005 unitamente alle opere sostitutive di passaggi a livello ricadenti nei Comuni di San Sostene e Badolato. Con nota del 29 luglio 2005, l'Amministrazione comunale, al fine di consentire l'attraversamento della linea durante l'esecuzione dei lavori, ha chiesto che l'inizio dei lavori fosse subordinato all'istituzione di un nuovo passaggio a livello provvisorio adiacente a quello esistente. La richiesta di variazione comporta, oltre ad un aumento dei costi, anche la realizzazione di una nuova intersezione stradale sulla strada statale 106 e, quindi, la necessità di una rielaborazione del progetto e l'attivazione delle procedure per l'ottenimento del benestare di competenza dell'ANAS di Catanzaro. E' da segnalare, peraltro, che le aree sono state formalmente consegnate dal Comune in data 11 maggio 2006. Dopo una prima riunione, tenutasi il 16 gennaio 2007, in cui è stato espresso parere favorevole alla realizzazione del sottovia, previa integrazione degli elaborati tecnici, l'ufficio ANAS competente ha rilasciato parere tecnico favorevole il 3 aprile 2007. In attesa della formalizzazione di tale parere, RFI sta procedendo, d'intesa con i tecnici ANAS, all'avvio dei lavori. Solo dopo l'attivazione del passaggio a livello provvisorio sarà possibile dare inizio ai lavori per la realizzazione del sottovia, che si prevede di completare nel maggio del 2008.

è testimonianza tipica della storia italiana: per fare un sottopasso occorrono venti anni. Credo che questo la dica lunga della situazione nella quale ci si trova. Ovviamente vengono attribuiti ritardi da un lato e dall'altro: all'Amministrazione comunale negli anni Ottanta e nei primi anni Novanta, adesso che la nuova Amministrazione comunale si è messa in moto per la rapida realizzazione di quest'opera si incontrano ritardi burocratici per quanto riguarda l'ANAS e le altre organizzazioni interessate. Tutto ciò

rende difficile procedere verso la modernizzazione e l'efficienza della nostra rete infrastrutturale, in modo particolare per quanto riguarda la messa in sicurezza delle aree

presa in giro nei confronti della popolazione, che attende da tempo che si metta in sicurezza quell'area e si eviti l'imbuto

le infrastrutture*. Si precisa che l'intervento relativo al lotto IV, oggetto dell'interrogazione, non è in fase di realizzazione da parte dell'ASI della Provincia di Avellino, bensì trattasi di progetto definitivo presentato dalla stessa ASI, in qualità di soggetto aggiudicatore, al Ministero delle infrastrutture in data 26 ottobre 2005 per le procedure approvative di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 190 del 2002, così come modificato dagli articoli 166 e 167 del decreto legislativo n. 163 del 2006. L'opera è inserita nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con delibera n. 121 del 2001, e nell'Intesa generale quadro sottoscritta in data 31 ottobre 2002 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la stessa Regione: collegamento autostradale Caserta-Benevento e Bretella di collegamento con l'autostrada Al (Caianello-innesto strada statale 372 "Telesina") e con l'autostrada A16 (Pianodordine-innesto raccordo Salerno-Avellino). Il progetto definitivo rappresenta un'evoluzione progettuale del progetto originario, al quale fa riferimento l'interrogante, nel tentativo di superare le evidenti difficoltà rappresentate dalla natura del terreno dal punto di vista geologico, per cui la progettazione definitiva ha tenuto conto, per quanto possibile, delle osservazioni espresse dalle varie amministrazioni e dai soggetti titolari dei sottoservizi e delle interferenze durante le Conferenze di servizi, indette dall'ASI, preliminari all'attivazione delle procedure approvative della cosiddetta legge obiettivo. Dette procedure hanno previsto la Conferenza dei servizi, indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi degli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 190 del 2002, durante la quale sono stati acquisiti pareri e proposte migliorative da parte dei soggetti interessati. Con riferimento ai pareri espressi dalle amministrazioni, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, si evidenzia che la Regione Campania, con delibera di giunta regionale del 15 marzo 2006, n. 340, ha espresso parere favorevole ai fini dell'intesa sulla localizzazione e parere favorevole sulla compatibilità ambientale

per le quali la procedura di VIA o la verifica risulta di competenza regionale, così come confermato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con propria nota del 10 novembre 2005, indirizzata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Relativamente al parere di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, la direzione generale regionale del medesimo Dicastero, con propria nota n. 10369 del 31 comunica di ritenere il progetto necessario di un approfondimento progettuale che affronti gli aspetti della mitigazione ambientale, relativamente alle problematiche di carattere naturalistico ricadenti sul territorio, con particolare riferimento alla richiesta di ridurre i lunghissimi viadotti ed i numerosi attraversamenti del fiume Sabato, nonché di una serie di indagini geoarcheologiche per l'intero tratto. Allo stato il soggetto aggiudicatore sta svolgendo le opportune attività di studio e analisi richieste. Assicuro il senatore interrogante che queste attività verranno attentamente monitorate

Questa sua apertura finale dimostra che erano fondate le ragioni della protesta del comitato locale, di molti cittadini e, aggiungo, della nostra interrogazione che - secondo motivo di apprezzamento

che, indipendentemente dai poteri del Parlamento e del Ministero, non si può non affrontare. Prima domanda: è realmente prioritario questo tracciato del progetto definitivo del IV lotto della Valle Caudina-Pianodardine? Io penso di no!

recente proposta, spero positivamente affrontata, della Napoli-Bari. Leggo sul quotidiano «Il Mattino» di ieri: «Grandi opere. Piano da 10 miliardi». Ancora si propone questo asse per 154 milioni di euro

al progetto definitivo senza aver valutato attentamente quello originario che lei cita? Non mi convincono le motivazioni addotte dagli uffici. C'è un problema geologico? Io posso documentare l'esatto contrario. Quella area è classificata come

Infine, è stata enormemente limitata la possibilità di accesso agli atti del comitato e lo strumento dell'interrogazione parlamentare è servito anche a fare emergere una serie di problemi. Io la invito realmente valutare in primo luogo quale sia il nesso con la legge obiettivo. Forse per spiegare

Non ho il tempo per descriverlo, ma è un progetto che lambiva i paesi e che evitava un impatto ambientale drammatico in un'area sia di enorme valore ambientale sia anche di enorme fragilità.

concertazione con le popolazioni locali. Uno dei punti all'ordine del giorno dell'Unione prevede che opere ad alto impatto ambientale vengano discusse con le popolazioni. Invito dunque il Governo e il suo Ministero a contattare la Regione Campania e la Provincia di Avellino perché si apra oltre che

L'interrogazione presentata dal senatore Davico, al di là della specifica questione rilevata attinente ai lavori in corso sull'autostrada Asti-Cuneo, consente di aprire una finestra sul complesso delle attività del Governo sull'intero settore delle concessioni autostradali. Le azioni del Governo hanno riguardato in modo incisivo l'universo della viabilità di interesse nazionale che, inserita nell'ambito dei corridoi europei e nella programmazione delle piattaforme produttive nazionali, deve anche essere opportunamente gestita per costituire un reale elemento di sviluppo. Si è agito su più livelli: in primo luogo, con la legge finanziaria 2007, si è previsto di stipulare con l'ANAS una nuova «convenzione unica», attualmente in corso di definizione, che rafforza i poteri di indirizzo pubblici nelle azioni della società. Essa sarà accompagnata da un piano economico finanziario di lungo periodo che definisca obiettivi e strategie aziendali e con una programmazione di breve periodo, cinque anni contro i tre precedenti, che consenta una ragionevole articolazione temporale di tale strategia. È stata data particolare importanza al settore autostradale che, come noto, è in grado di realizzare notevoli investimenti extra bilancio dello Stato in infrastrutture strategiche grazie alle tariffe riscosse dagli utenti. Anche in questo caso le nuove normative introdotte dal Governo mirano a rafforzare gli aspetti di pubblico interesse dell'istituto concessorio per garantire sia l'effettiva realizzazione delle infrastrutture previste nei piani finanziari, che sono risultate sistematicamente in ritardo, che a riequilibrare a vantaggio degli utenti le regole tariffarie del settore, evitando ingiustificati profitti nel caso di mancata realizzazione degli investimenti. Un primo intervento normativo sul settore, di carattere quasi emergenziale, comprendente anche regole assicuranti una migliore trasparenza nelle gestioni ed una maggiore concorrenza nell'esercizio delle attività concesse, è intervenuto con il decreto legge n. 262 del 2006, convertito nella legge n. 286 del 2006, introducendo l'obbligo di inserire tali nuove regole in una nuova convenzione unica da stipularsi tra ANAS e tutte le concessionarie autostradali. La manovra è stata perfezionata con la legge finanziaria, precisando ulteriormente tali nuove regole e i derivanti aspetti operativi. I criteri di tali norme sono stati recepiti sotto il profilo tecnico dalla delibera CIPE n. 1 del 26 gennaio 2007. Delineato il quadro normativo, si è passati al piano operativo applicativo, pervenendo rapidamente alla definizione concordata della «convenzione unica» con sei concessionari autostradali. Altresì, in occasione della definizione delle tariffe annuali 2007 dei concessionari autostradali, si è superato l'aggiornamento automatico, determinando il livello tariffario in funzione degli investimenti realizzati. In particolare tra i mesi di marzo ed i primi giorni di maggio si è pervenuti a concordare l'intesa sulle nuove regole convenzionali con sei concessionari (BREBEMI il 26 marzo 2007; Pedemontana Lombarda il 20 aprile 2007; Asti Cuneo il 7 maggio 2007; Brescia Padova, Venezia Padova, Autocamionale Cisa l'8 maggio 2007); i testi concordati con le concessionarie hanno iniziato l'*iter* approvativo previsto dall'articolo 2, comma 84, delle legge n. 286 del 2006, come modificato dal comma 1030 della finanziaria 2007. Complessivamente le convenzioni uniche in parola consentono di avviare investimenti per circa complessivamente 11.471 milioni di euro, a prevalente carico di risorse extra bilancio dello Stato, con effetti positivi sul PIL e con l'avvio a soluzione di alcune delle più grandi criticità infrastrutturali presenti nelle zone più produttive e congestionate del Paese, ma con benefici effetti sull'intero sistema Paese. Tra le opere più rilevanti oggetto delle convenzioni così rinnovate, è incluso il completamento del collegamento autostradale tra Asti e Cuneo, che risolve un sentito problema locale di isolamento dalle grandi vie di comunicazione. Il 7 maggio è stato difatti siglato a Torino lo schema di convenzione tra ANAS e la società concessionaria per la realizzazione degli ultimi lotti di completamento dell'autostrada e per la gestione dell'intera rete autostradale. Lo schema di convenzione, elaborato in conformità alla recente normativa sulle concessioni autostradali, seguirà l'*iter* approvativo disposto dalla legge, che prevede la trasmissione al CIPE, il parere del NARS e delle competenti Commissioni parlamentari, e l'emanazione del decreto interministeriale di approvazione del testo finale della convenzione. All'esito, la società concessionaria potrà avviare i cantieri sui rimanenti 53 chilometri di autostrada, i cui tempi di realizzazione sono previsti in quattro anni, con ultimazione dei lavori tra il 2010 e il 2011. Lo schema di convenzione ha anche fissato il cronoprogramma dei lavori. ANAS vigilerà sul rispetto dei tempi e sulla qualità dei progetti e dei lavori. Tanto premesso in linea generale, si risponde allo specifico quesito posto nell'interrogazione inerente la situazione sulla tratta autostradale Asti-Cuneo in conseguenza del sequestro del Lotto tra Isola d'Asti e Motta di Castigliole disposto dall'autorità giudiziaria lo scorso 27 marzo. In merito, si informa che la procura della Repubblica presso il tribunale di Asti ha disposto in data 6 aprile il dissequestro del tratto autostradale essendo venute meno le esigenze istruttorie alla base del provvedimento e venendo così incontro alle richieste di ANAS nella qualità di parte offesa. Il lotto in questione è stato quindi inaugurato ed aperto al traffico il 16 aprile contestualmente agli altri lotti (Motta-Covone e Covone Neive Guarene). I necessari lavori di ripristino della pavimentazione stradale, male eseguita per circa 1,3 chilometri, saranno effettuati a carico dell'impresa in soggezione di traffico. L'ANAS ha assicurato sin dall'inizio della vicenda la massima collaborazione alla magistratura, garantendo l'assoluta sicurezza di guida e il proprio impegno ad eseguire i lavori di risanamento della pavimentazione, nel minor tempo possibile e con il minimo disagio per l'utenza. Ciò ha consentito, come detto, di aprire al traffico, nei tempi previsti, 18 nuovi chilometri dell'autostrada Asti-Cuneo, tra Isola d'Asti e Alba, nonché la nuova variante di Isola d'Asti. I tre lotti aperti consentono un collegamento diretto tra Isola d'Asti e Alba, decongestionando la viabilità nei centri di Castigliole, Covone, Magliano Alfieri, Castagneto e Guarente. Per quanto riguarda i lotti di diretta competenza ANAS, entro giugno 2007 saranno aperti al traffico gli ultimi due lotti ANAS e cioè il Lotto 7 (Diga ENEL-Cherasco) e il Lotto 8 (Cherasco-Marene) in concomitanza con l'ultimazione dei lavori di costruzione del casello di Cherasco. Pertanto, entro tale data saranno aperti al traffico 37,5 chilometri di autostrada su un totale di 90,5 chilometri,

questa interrogazione, come lei ben dice, permette di fare qualche ragionamento che va oltre ciò che è successo, che chiaramente

sono tratti neppure collegati tra loro e creeranno nella viabilità collaterale non pochi problemi, non poche conseguenze, non poche difficoltà, anzi andranno ad appesantire e a determinare

quando, a seguito delle irrevocabili dimissioni presentate dal Sindaco, il prefetto di Avellino ha proceduto a norma di legge a sospendere il Consiglio comunale di Sant'Angelo dei Lombardi ed a nominare un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente,

Quanto alla situazione specificatamente segnalata nell'interrogazione, dalle notizie riferite dalla prefettura di Avellino risulta che, in occasione delle elezioni amministrative del 12 e 13 giugno 2004, nel Comune di Sant'Angelo dei Lombardi furono presentate due liste civiche che candidavano alla carica di Sindaco rispettivamente il primo cittadino uscente, Antonio Petito, e la figlia di quest'ultimo, Lucia Petito in Guerriero. Verosimilmente, come evidenziato anche dal senatore Tecce, la lista «Unione e Progresso», capeggiata dalla signora Petito, fu presentata per scongiurare il verificarsi dell'ipotesi di cui all'articolo 60 del decreto del che, nei Comuni inferiori a 10.000 abitanti, come noto, in caso di presentazione di una sola lista di candidati, richiede per la validità delle elezioni la partecipazione al voto di non meno del 50 per cento degli aventi diritto. L'ipotesi che si trattasse di una cosiddetta lista civetta è suffragata dal fatto che l'altra formazione, capeggiata dal Sindaco uscente, riportò poi una percentuale di suffragi pari al 95,8 per cento, a conferma dell'assenza di una reale competizione fra i candidati. Successivamente, perveniva all'autorità giudiziaria una denuncia con la quale un uomo ammetteva di aver falsificato la sottoscrizione di accettazione della candidatura nella lista civetta da parte della propria consorte grazie alla compiacenza dello stesso Sindaco uscente. A seguito di tale chiamata in correità, il GIP presso il tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in data 14 maggio 2005, emetteva decreto penale di condanna nei confronti del Petito, comminandogli un'ammenda di 700 euro con beneficio della sospensione condizionale per aver concorso nel reato previsto dall'articolo 90, terzo comma, del decreto del come modificato dalla legge n. 61 del 2004 in relazione all'articolo 476 del codice penale, che punisce chiunque commetta un reato di falso in merito all'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero formi falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati. In particolare, al Petito fu contestato di aver autenticato, nelle sue funzioni di pubblico ufficiale in quanto Sindaco del Comune, la firma falsa apposta dal marito a nome della moglie. Analogo reato è stato contestato anche in relazione all'autenticazione dì altra firma falsa apposta da un terzo coimputato. Avverso il decreto penale di condanna, l'interessato proponeva opposizione ed il relativo procedimento risulta ancora pendente, con udienza fissata davanti al giudice monocratico per il 27 giugno prossimo. Nel valutare la situazione venutasi a determinare in seguito al pronunciamento emesso con decreto penale di condanna (che non è ancora divenuto definitivo), il prefetto di Avellino ritenne che, non essendovi alcun provvedimento di annullamento delle operazioni elettorali emesso in sede giurisdizionale, il Consiglio comunale dovesse rimanere in carica, non sembrando ricorrere alcuna delle ipotesi di scioglimento del consesso elencate e previste dalla legge. Tale orientamento veniva condiviso dagli uffici del Ministero dell'interno che il 26 maggio 2005, rispondendo ad un quesito del prefetto di Avellino, rilevava come non fosse applicabile il combinato disposto degli articoli 58 e 59 del citato Testo unico sugli enti locali. Tali norme, infatti, prevedono la decadenza di coloro i quali, dopo aver assunto la carica, siano colpiti da una condanna definitiva per il reato in essi elencati, fra i quali non figura quello contestato al signor Petito, o comunque per un reato commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione a condizione che vi sia stata condanna ad almeno sei mesi di reclusione, laddove invece nel caso di specie era stata comminata solo una pena pecuniaria. Quanto alla surroga di un consigliere dimissionario con una persona la cui accettazione di candidatura è risultata falsa in sede penale, sollevata dall'interrogante, la prefettura di Avellino ha ritenuto decisivo il fatto che l'interessata non abbia mai impugnato né il provvedimento della commissione elettorale circondariale di ammissione della candidatura della lista civetta ove la stessa era inserita né le conseguenti operazioni di voto. Si è così determinata una situazione che, convengo con l'interrogante, presentava indubbiamente dei profili sostanziali molto dubbi e che tuttavia, come ho già detto, è venuta meno con il già citato provvedimento di sospensione prima e di scioglimento poi del Consiglio. Ritengo peraltro che il caso evidenziato dal senatore Tecce si sia potuto verificare a causa di una non perfetta coerenza di talune disposizioni dell'ordinamento degli enti locali con le norme sul procedimento elettorale; problema certamente rilevante che potrà eventualmente essere valutato in sede di esame del disegno di legge delega per la nuova Carta delle autonomie locali, attualmente in discussione proprio presso questo ramo del Parlamento.

e per gli spunti di riflessione che ci offre. Ovviamente, come lei ha riscontrato, l'oggetto dell'interrogazione è già superato. Il Consiglio comunale di Sant'Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino è stato sciolto. La cronistoria che lei ha fatto integra e rafforza, dal mio punto di vista, la gravità dei reati che avevamo evidenziato.

insieme compiono un atto grave, ammesso da uno dei due, il Del Goleto, con un'autodenuncia: come spesso avviene in questi paesi, prima fanno la lista assieme e poi litigano per motivi politici o presunti tali.

legge. Un'altra riflessione molto positiva mi viene dalla sua risposta: il valore - lo dico a lei, presidente Baccini - del sindacato ispettivo e della funzione di controllo del Ministero dell'interno sugli enti locali.

regionali crei qualche problema. In ogni caso, il dato positivo è che la presentazione dell'interrogazione, l'attività del prefetto che lei cita, con la richiesta dei quesiti, e l'iniziativa di mobilitazione della popolazione hanno portato all'autoscioglimento, perché, man mano che le persone venivano cooptate, qualcuno ha avuto paura e si è dimesso, per cui si è sciolto il Consiglio comunale. Un'ultima riflessione. Lei lo ha detto, al di là degli aspetti formali, il profilo sostanziale è che una lista prende il prende quanto è fisiologico. Noi dobbiamo riflettere sulla normativa, resa al Sud più delicata per il fatto che molte liste elettorali sono piene di persone emigrate in Argentina e in Venezuela

rispondo all'interrogazione del senatore Gramazio riguardante le modalità di controllo del territorio e di vigilanza a fini di prevenzione generale attuate sul territorio della città di Roma. Premetto innanzi tutto che le politiche in atto in materia di sicurezza tendono ad un generale obiettivo dì maggiore efficienza ed efficacia dell'attività delle Forze di polizia, da perseguire anche attraverso una complessiva razionalizzazione e riorganizzazione, volta ad ottimizzare il rapporto fra risorse impiegate e risultati ottenuti. In questa direzione si muovono, da ultimo, talune norme contenute nell'ultima legge finanziaria. È il caso dell'articolo 1, comma 439, della legge n. 296 del 2006, che prevede la possibilità di stipulare convenzioni con le Regioni e gli enti locali per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, ovvero dei commi 431 e 435 dello stesso articolo, relativi rispettivamente alla razionalizzazione delle strutture di supporto dell'amministrazione della pubblica sicurezza ed alla predisposizione di appositi piani pluriennali di riarticolazione e ridislocazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia, entrambi in funzione di una razionalizzazione delle spese correnti che consenta una più oculata ed efficace destinazione delle risorse. L'obiettivo è il reimpiego ottimale delle risorse umane, logistiche, tecnologiche e strumentali finalizzato ad un incremento dell'efficienza del sistema di sicurezza territoriale, con una contestuale riduzione di spese correnti per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio, almeno pari al 5 per cento entro il 2007 e ad un ulteriore 5 per cento entro il 2008. Ad analoghi fini di buona amministrazione ed ottimizzazione delle risorse si ispirano anche provvedimenti assunti localmente, come la rimodulazione degli orari di servizio di alcuni commissariati di Roma, cui fa cenno l'interrogante e di cui dirò fra poco. Tengo tuttavia a sottolineare subito come non vi sia stato alcun depotenziamento dell'attività delle volanti sul territorio di Roma. Negli ultimi due anni, il reparto volanti ha mantenuto costante una presenza media di 13-14 pattuglie per ogni quadrante orario, per un totale complessivo di 52-54 volanti ai giorno, cui si aggiungono le 32 autoradio per quadrante dei commissariati di polizia, per un totale di 128 al giorno. Pertanto, nell'arco complessivo di un'intera giornata, le unità operative presenti sul territorio sono circa 180, cui, fra le 8 e le 20, ne vanno sommate almeno altre quattro dedicate all'attività di contrasto del fenomeno delle rapine aggravate nell'ambito di competenza dei commissariati Aurelio, Monteverde, San Paolo e San Basilio. La rimodulazione degli orari di servizio dei commissariati, infatti, non intende certo ridurre lo sforzo profuso nell'attività di controllo del territorio, tanto meno sottende una valutazione sul fatto che alcuni quartieri siano più tranquilli di altri. Tutt'altro: i servizi erano e rimangono capillarmente distribuiti su tutto il territorio cittadino, benché adattati e modellati sulle specifiche caratteristiche di ciascuna area. In quest'ottica, coerentemente con i princìpi generali di riorganizzazione degli impieghi di mezzi e personale, si è però cercato di utilizzare al meglio le risorse e di indirizzarne miratamente una parte proprio verso il contrasto e la prevenzione di quelle specifiche fattispecie predatorie, come le rapine agli esercizi commerciali ad alto afflusso di pubblico, richiamate nell'interrogazione. In particolare, l'aver concentrato in una fascia oraria più ristretta (dalle 8 alle 20) le pattuglie di quattro commissariati fra loro non contigui ha consentito di triplicare la presenza delle unità operative nelle ore più critiche, dando anche un'ulteriore, concreta risposta alle aspettative dei commercianti e dei residenti. Il pattugliamento notturno viene invece assicurato attraverso la pianificazione dell'attività coordinata di diverse unità della sezione volanti e dei commissariati tra loro vicini, che continuano ad applicare un orario articolato su quattro turni (07-13, 13-19, 19-24, 24-07), senza alcuna variazione rispetto al passato. In tal modo, si è realizzato un aumento del 6,6 per cento delle unità dei commissariati sezionali addette al controllo del territorio. Il provvedimento di rimodulazione oraria si inserisce in un più ampio ed organico complesso di misure, che vanno dalla sorveglianza mirata dei soggetti maggiormente pericolosi a un più intenso raccordo delle attività investigative, secondo un preciso disegno anticrimine che trova conforto sia nell'incremento delle unità utilizzabili, sia, nelle zone interessate, in un primo ridimensionamento del fenomeno che si intendeva contrastare più efficacemente. A tal proposito, si soggiunge che, dall'analisi dei dati sull'attività di prevenzione in città, si registra un incremento dei controlli tanto nei confronti di persone

sia dell'intensità e capillarità dei dispositivi di controllo in atto sul territorio metropolitano, la cui pianificazione e programmazione si presenta idonea a consentire un efficace perseguimento delle esigenze di sicurezza presenti nella città di Roma.

i sindacati di categoria della Polizia di Stato hanno tenuto a Roma una conferenza stampa che riprendeva in parte la mia interrogazione a proposito della riduzione dei mezzi della Polizia di Stato che escono dalla caserma di Via Guido Reni: la sera ne uscivano 30, mentre adesso ne escono 10. Queste sono verità, sono verità, riportate ampiamente dai funzionari della Polizia di Stato che hanno partecipato a tale conferenza stampa sui temi della criminalità organizzata nella città di Roma.

nelle strade dei singoli quartieri. Vorrei richiamare alla sua attenzione, ma sicuramente lei ne ha a conoscenza, che a volte è molto meglio una macchina visibile della Polizia di Stato, dei Carabinieri o della Guardia di finanza, perché queste, passando in una strada commerciale, evitano il borseggio.

poiché ormai tutti i supermercati, specialmente nelle zone che ho richiamato nella mia interrogazione, hanno bisogno di protezione, perché si svolgono rapine quasi quotidiane. Quindi, mi auguro una maggiore attenzione da parte del Ministero dell'interno per la città di Roma

I fatti cui si riferisce l'interrogazione si sono verificati il 5 marzo scorso a Roma, quando circa 300 persone aderenti a Action, Comitato lotta per la casa e Comitato obiettivo casa, hanno inscenato presso il Campidoglio un'estemporanea manifestazione di protesta per sollecitare il Comune alla soluzione di alcune problematiche abitative. Durante la manifestazione, due giovani hanno invocato, uno dopo l'altro, l'intervento delle Forze dell'ordine, denunciando di essere stati oggetto di aggressione fisica o verbale da parte di alcuni manifestanti. Il primo riferiva di essere stato minacciato e apostrofato come fascista da alcuni manifestanti, mentre con alcuni coetanei si accingeva a recarsi alla seduta del Consiglio comunale al seguito del consigliere di Alleanza Nazionale Federico Guidi. Il secondo, che presentava una leggera tumefazione al labbro inferiore, dichiarava di essere stato malmenato mentre tentava di raggiungere lo stesso consigliere Guidi, rifiutandosi peraltro di sporgere denuncia e di ricorrere al soccorso medico. In relazione ai fatti, la Polizia di Stato ha segnalato all'autorità giudiziaria, in stato di libertà, 37 persone per avere promosso, in violazione dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, una manifestazione pubblica senza averne dato preavviso al questore. A causa della rapidità degli eventi, non è stato viceversa possibile identificare con immediatezza gli autori dell'aggressione compiuta ai danni dei giovani esponenti di Alleanza Nazionale; sono comunque in corso indagini tese alla loro individuazione. Al momento, non risulta peraltro presentata alcuna querela di parte per gli episodi in questione. Per quanto riguarda il quesito sulle iniziative intraprese per evitare il ripetersi di atti di intolleranza ai danni dei consiglieri comunali, preciso che le autorità di pubblica sicurezza e le Forze di polizia seguono con la massima attenzione tutti gli eventi che incidono negativamente sulla sicurezza e sulla libertà di espressione degli amministratori e degli esponenti delle forze politiche. Il Ministero dell'interno sta svolgendo, a tal fine, un'attenta opera di impulso e sensibilizzazione delle questure per l'intensificazione delle strategie di contrasto e l'adozione di mirati moduli operativi. A tal fine, dopo l'episodio richiamato dal senatore Gramazio, è stata ulteriormente raccomandata agli uffici di Polizia una ancora più attenta vigilanza degli obiettivi esposti a rischio. Preciso, al riguardo, che la vigilanza delle sedi di partiti, circoli, movimenti politici e organizzazioni sindacali, così come, quando necessario, la protezione degli amministratori locali e di tutte le persone esposte a rischio a causa delle funzioni esercitate, costituisce una delle priorità nella pianificazione dei servizi di controllo del territorio svolti dalle Forze dell'ordine in ogni regione del Paese, secondo una programmazione definita Provincia per Provincia. II Ministero dell'interno non sottovaluta, quindi, la gravità ed il significato di nessun episodio di violenza o intolleranza politica, neppure quelli più estemporanei, occasionali e non preordinati, in quanto comunque espressione del riaffiorare di una tendenza a condizionare con la violenza la normale dialettica democratica. L'esigenza di prevenirne il ripetersi in occasione di eventi e pubbliche manifestazioni viene attentamente considerata anche in sede di predisposizione dei relativi servizi di ordine pubblico, attraverso l'adozione di misure finalizzate a ridurre o minimizzare le occasioni di contatto e contrapposizione

due ragazzi giovanissimi, i quali, proprio per la loro età, non si sono voluti nemmeno fare ricoverare presso il pronto soccorso della città e non hanno voluto sporgere denuncia per non intimorire i propri genitori per l'aggressione subita. Ho voluto evidenziare questo aspetto proprio perché ritengo necessaria, gentile Sottosegretario, l'attenzione da lei

presentata al Ministro dell'ambiente, in ordine a presunti pagamenti effettuati dal commissario per l'emergenza ambientale nella Regione Calabria per 41 unità assunte con contratti stipulati direttamente a Roma dai dirigenti del Ministero dell'ambiente che sembrerebbe non abbiano mai partecipato alle attività dell'ufficio del commissario stesso. Nel frattempo, dalla presentazione dell'interrogazione ad oggi, il commissario è cambiato - è l'ottavo - e c'è un altro prefetto.

il problema di 110 aziende che lavorano con il Servizio sanitario regionale, dunque fornitrici di beni e servizi alla Regione Lazio, alle ASL e alle aziende ospedaliere, che versano in gravi difficoltà